«Il Presidente della Repubblica, VISTO l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; CONSIDERATA la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 settembre 2009, recandosi nella Repubblica di Corea in visita di Stato ed in Giappone in visita ufficiale; DECRETA: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 settembre 2009 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 2009 *Firmato*Giorgio Napolitano *Controfirmato*Silvio Berlusconi». In conseguenza della situazione costituzionale così determinatasi, la vice presidente del Senato Rosa Angela Mauro è stata incaricata di esercitare per tutto il periodo della supplenza le funzioni di Presidente del Senato in base alla designazione effettuata in data 23 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento. Onorevoli colleghi, nella giornata di ieri, dopo aver appreso che il senatore Massimo Livi Bacci è stato aggredito a Firenze da due malviventi che lo hanno rapinato e colpito al volto, ho immediatamente manifestato al nostro stimato collega i sentimenti di vicinanza e solidarietà miei personali e di tutta l'Assemblea. Nel condannare fermamente la vile aggressione e nell'auspicio che i colpevoli di questa azione violenta e insensata siano assicurati al più presto alla giustizia, desidero rinnovare al senatore Livi Bacci i più affettuosi auguri di pronto ristabilimento da parte di tutti la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, nel confermare il calendario della settimana corrente ha approvato il calendario della prossima settimana fino a giovedì 24 settembre. A partire dalla seduta pomeridiana di martedì 22 settembre sarà discusso il decreto-legge recante disposizioni correttive del decreto anticrisi, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Gli altri argomenti da esaminare nel corso della prossima settimana, anche sulla base dei solleciti dei Gruppi, saranno definiti dalla Conferenza dei Capigruppo, che sarà convocata nella giornata di martedì 22 settembre, con particolare riguardo alle mozioni sul Fondo aree sottoutilizzate. Nel corso di tale riunione sarà inoltre discussa la questione nuovamente posta dal Gruppo dell'Italia dei Valori circa la mancata presenza di un proprio rappresentante nel Consiglio di Presidenza.

per quel che riteniamo essere un *vulnus* che si è originato oltre un anno fa e al quale, nonostante le parole

Per quella che possiamo definire una manovra non proprio limpida, per usare un eufemismo, vi è stato un incrocio di voti e di volontà - speriamo solo di voti e non anche di volontà - che ha portato all'esclusione dell'Italia dei Valori dal Consiglio di Presidenza. del ruolo che tutti i Gruppi, anche quelli che sono sottogruppi all'interno di Gruppi, hanno all'interno dell'Assemblea, a noi pare vergognoso di un Gruppo che rispetta le regole del gioco, collabora all'attività di formazione delle leggi e manifesta un interesse a risolvere i problemi del Paese, ovviamente dal proprio punto di vista politico, venga adottata una *conventio ad excludendum* che non è motivata né dalla forza elettorale del Gruppo né dal lavoro che il Gruppo stesso fa nelle Commissioni e in Aula, dove cioè si esplica l'attività costituzionalmente riservata al Parlamento.

dar corso oggi ad ulteriori gesti eclatanti, manifestiamo all'Assemblea la nostra ferma volontà di non muoverci

non siamo presenti nel consiglio di amministrazione che gestisce la società Senato. Ovviamente ho ragionato per metafora e non certamente perché perché consideri il Senato una SpA, proprio per rendere più evidente il senso delle mie parole. Quindi, intendiamo mantenere questo presidio simbolico e visibile, ma diciamo all'Assemblea e alla Presidenza che non riteniamo esaurita questa forma di protesta fino a quando il problema non sarà realmente risolto.

martedì prossimo con il presidente Schifani - affrontare questo problema per arrivare ad una soluzione che possa accontentare tutti. Riteniamo però sbagliato il modo con cui oggi si vuole presentare questa richiesta dal Gruppo dell'Italia dei Valori. L'impressione, colleghi dell'Italia dei Valori, che potete dare al di fuori di quest'Aula è che qui c'è un Parlamento che ha voglia di lavorare e voi invece siete in questo Parlamento per occupare dei posti che non sono vostri in questo momento. *(Commenti del senatore Astore)*. I senatori Segretari d'Aula sono stati eletti da questa Assemblea,

scrutinio segreto dell'Aula sono state chiare, solari e rispettose delle facoltà e dei diritti di ognuno, nonostante le modalità di protesta difficilmente accettabili che anche oggi il Gruppo dell'Italia dei Valori ha scelto

completa, possa consentire all'Italia dei Valori di riprendere i lavori di questa seduta in modo ordinario e quindi, se non di cessare, almeno di sospendere momentaneamente la protesta in atto.

Presidente, chiedo che la seduta venga sospesa per dieci minuti.

Presidente, così come l'occupazione simbolica

considerata un ricatto né una pressione, così la disponibilità a far continuare regolarmente i lavori non deve essere intesa come un segnale di debolezza o di arretramento di fronte ad una posizione severa che abbiamo assunto. assunto. Noi prendiamo atto pertanto - l'ho già anticipato - di una disponibilità sostanziale, peraltro già manifestata più volte, e interrompiamo questa forma di protesta senza che ciò venga inteso in modo diverso da quello che è, perché non ci sono né retropensieri né altro.

Il nostro *bon ton*, il nostro buon senso e la nostra pazienza - ripeto - non possono essere intesi come una sorta - permettetemi il termine alla latina

il testo che oggi viene sottoposto all'approvazione della nostra Assemblea trae origine dal lavoro di approfondimento compiuto nella presente legislatura

La questione del furto di identità e della protezione dei consumatori e degli operatori nell'ambito delle attività che prevedono il pagamento differito ha assunto infatti dimensioni di grande rilevanza. L'incremento del ricorso allo strumento del credito al consumo e ai pagamenti dilazionati o differiti da parte di persone fisiche e giuridiche ha determinato una crescita esponenziale del numero delle frodi nel settore dei finanziamenti, tale da creare un giustificato allarme per le conseguenze negative. La Banca d'Italia, nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, riceve dagli operatori informazioni statistiche sulle operazioni di pagamento e prelievo di contante per il tramite di carte di credito per le quali si sono verificate frodi. Dai dati disponibili si desume che il fenomeno delle frodi attraverso questi strumenti di pagamento è rilevante: in particolare, tra il 2004 e il 2006 esse sono risultate in costante ascesa, sia in termini di importo complessivo

Il furto di identità, cioè la sottrazione di dati personali dell'interessato, è un fenomeno in crescita preoccupante, che comporta per le vittime costi economici e psicologici sempre più alti.

Se poteste rispettare l'intervento della relatrice senza costringere la Presidenza a vari richiami credo ne gioverebbe il dibattito oltre che Sono diversi i modi in cui i frodatori si procurano illegalmente i dati personali. Tra i più diffusi in ambito informatico c'è sicuramente il *phishing*, frode attraverso la quale vengono richiesti ed acquisiti illegittimamente i dati personali di soggetti, in genere tramite *e-mail*, simulando un'istituzione nota al destinatario, per esempio la sua banca, o il più recente *pharming*, tecnica attraverso la quale gli *hacker* riescono con sofisticate tecniche di intrusione a manipolare le direzioni verso le quali viaggiano le informazioni relative agli indirizzi *web*. Quindi, ad esempio, digitando l'indirizzo Internet della propria banca, l'utente viene reindirizzato, senza accorgersene, su un sito creato dal *pharmer*. Dai dati di una recente indagine condotta da ABI ed ASSOFIN su un campione di operatori, che dà conto dell'elevato costo del fenomeno e del suo accentuarsi estremamente pericoloso, è emerso che il danno per i consumatori si verifica a tre livelli: il primo è quello della maggiore difficoltà ad ottenere il credito, il secondo è rappresentato dall'impatto il terzo è quello dei costi che il consumatore sostiene quando la sua identità è utilizzata da terzi per ottenere finanziamenti che non vengono, ovviamente, rimborsati.

cioè poche settimane prima che esplodesse una delle più grandi tempeste finanziarie del secolo, con il fallimento di Lehman Brothers. Quel giorno la moglie di Bernanke, Anna, subì il furto della borsetta contenente, tra l'altro, patente, tessera della *Social Security*, carte di credito e un libretto di assegni. Il furto venne subito denunciato alla banca e alla polizia e ciò evitò al capo della FED di subire un danno finanziario.

che, mescolando metodi tradizionali all'uso delle più avanzate tecnologie, ripuliva i conti bancari di centinaia di persone.

Negli Stati Uniti, il Governo ha già varato una legge *ad hoc* per il furto di identità. In Europa, invece, per simili reati si applicano ancora leggi relative a vecchi reati, quali truffa, violazione della *privacy* e, a volte, produzione di falsi documenti. Solo recentemente il Movimento dei consumatori italiani ha depositato due denunce in materia: la prima riguardava lo scambio di identità,

Di fronte alla pericolosità sociale di questi fenomeni la Commissione europea ha subito preso un'iniziativa concreta, decidendo di disporre uno studio comparativo sulle singole leggi che possono riguardare il furto di identità. Lo studio dovrà quindi fornire una mappatura delle iniziative già esistenti o già pianificate, in modo da offrire alle vittime di questi furti gli strumenti più tempestivi per ottenere assistenza. Nel dettaglio, lo studio dovrà riguardare un'analisi delle specifiche legislazioni, esempi di come la legislazione viene applicata in ogni Paese (incluse le sanzioni), una revisione dei meccanismi di denuncia esistenti o pianificati che assistono le vittime di furti di identità negli Stati dell'Unione europea e nei Paesi terzi pertinenti in base ai meccanismi di denuncia identificati, le raccomandazioni su come promuovere la costituzione di sportelli unici per le vittime del furto di identità nell'Unione europea. Per venire al nostro Paese, secondo le stime del CRIF in Italia sono state realizzate 25.000 frodi per un importo di circa 145 milioni di euro relativi sono in continua espansione. Anche nel settore assicurativo le frodi esistono, al pari di quelle commesse negli altri settori finanziari, e comportano effetti rilevanti sulla collettività. però qualcosa di ancora più preoccupante, che riguarda la capacità da parte di siti illegali di offrire in vendita in modo aperto e plateale sul *web* i codici di accesso ad altre identità digitali: in una parola, si può comprare la *password* altrui alla modica cifra di 100 dollari. Proprio perché si tratta di un fenomeno in continua espansione occorre perseguire l'obiettivo - e così veniamo al testo dei disegni di legge in esame - di creare un modello di prevenzione e monitoraggio sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti puntando su tre direttrici: prevenire il fenomeno, attraverso strumenti di accertamento dell'identità e dell'effettiva capacità di reddito del soggetto che richiede il credito; costituire un deterrente in grado di dissuadere i potenziali frodatori; ridurre il contenzioso giudiziario in materia civile e penale. Il testo che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ha quindi origine, come dicevo prima, da un lungo e approfondito lavoro svolto in stretta collaborazione tra la Commissione, il Governo e gli organismi preposti alla vigilanza e al controllo su specifici settori, come la Banca d'Italia, l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali.

finanza. Il lavoro della relatrice è stato certamente facilitato dalla sostanziale omogeneità dei due disegni di legge presentati, nonché dalla circostanza di un'unitarietà di intenti tra i Gruppi che che ha reso possibile l'adozione di misure condivise. L'impianto della proposta legislativa riprende quindi quello dei disegni di legge dei senatori Barbolini e Costa e, per una descrizione analitica, si fa rinvio alle relazioni introduttive ai due testi originari. È utile rimarcare le novità introdotte rispetto a tali proposte, volte a migliorare il testo e a renderlo maggiormente aderente alle esigenze degli operatori. Va innanzitutto detto che il testo prevede, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare dell'archivio, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento ( UCAMP), l'istituzione di un sistema di prevenzione basato sull'archivio centrale informatizzato. Nel titolo e nel comma 1 dell'articolo 1 è stata inserita la specificazione che le finalità dell'intervento legislativo comprendono anche la prevenzione del furto d'identità e non soltanto, su un piano più generale, ma anche più generico, le frodi nel settore del credito al consumo e in quello assicurativo. Al comma 3 è stata inserita una clausola di salvaguardia dei poteri di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attribuzione all'UCAMP della titolarità dell'archivio e della responsabilità della gestione dello stesso. Al comma 4 si sono precisati maggiormente gli ambiti operativi nei quali si esercitano le competenze dell'UCAMP, operando anche un rinvio all'articolo 121 del testo unico bancario per la definizione della nozione di credito al consumo. Per quanto riguarda l'individuazione degli aderenti al sistema di prevenzione, si è ritenuto opportuno inserire, alla lettera *a)* del comma 5, le banche comunitarie stabilite nel territorio dello Stato, quelle extracomunitarie autorizzate a termini di legge, nonché gli intermediari finanziari non vigilati, cui all'articolo 106 del testo unico bancario. Sono state inserite due altre categorie di soggetti aderenti costituite dalle società di mediazione creditizia, precisando un requisito di capitale sociale minimo, e i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi. È stato inoltre previsto che le forze dell'ordine - Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato - possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi. Al comma 6 si è specificato che la verifica dell'autenticità dei dati è circoscritta ai casi e alle finalità di prevenzione e contrasto del furto d'identità. È stato anche sostituito il comma 7, prevedendo l'istituzione di un servizio telefonico e telematico per l'invio delle segnalazioni delle frodi subite configuranti ipotesi di furto d'identità. È stata ampliata la composizione del gruppo di lavoro, prevedendo prevedendo anche la partecipazione dei rappresentanti della Banca d'Italia, dell'ISVAP, delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti, degli operatori commerciali, delle associazioni dei consumatori e del Garante per la protezione dei dati personali. Si è inoltre stabilito di inserire nella relazione al Parlamento anche una specifica sezione con i risultati dell'attività di verifica del Garante e l'attribuzione all'UCAMP del compito di svolgere campagne informative sui rischi

costituito dal modulo di allerta, mentre in relazione al modulo informatico centralizzato è stata specificata la possibilità di predisporre e pubblicare periodicamente apposite linee guida sull'evoluzione del fenomeno delle frodi. È stata infine prevista la comunicazione dei risultati dell'attività di prevenzione dell'UCAMP al Ministero dell'interno e all'ISVAP per finalità di repressione e contrasto della criminalità Nell'articolo 3 si è precisato il novero delle informazioni oggetto di riscontro, introducendo alcune precisazioni di carattere lessicale, mentre è stato previsto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Garante per la protezione dei dati personali, il rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione per l'individuazione di eventuali ulteriori informazioni suscettibili di verifica. Nella prospettiva di garantire la tutela dei consumatori si è inserito un ulteriore comma all'articolo 4, che prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi per monitorare le variazioni delle condizioni economiche praticate dagli aderenti al sistema nei confronti dei consumatori. Sono state riformulate le disposizioni finanziarie in accoglimento del parere della Commissione bilancio, di cui all'articolo 5. L'articolo 6 contiene una norma di rinvio ad un decreto ministeriale per l'attuazione delle disposizioni, prevedendosi l'intervento del Parlamento, attraverso l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, oltre che della Banca d'Italia e del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 7, infine, contiene norme relative al sistema di prevenzione frodi nel settore assicurativo, senza particolari modifiche rispetto ai testi presentati in precedenza, con l'eccezione del parere dell'ISVAP e della clausola di salvaguardia finanziaria in assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Queste, brevemente, sono le novità rispetto ai disegni di legge originari. In conclusione, auspico un rapido *iter* del provvedimento in modo da consentire successivamente alla Camera dei deputati di avviarne celermente l'esame.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Leddi. Ne

si sottostima la portata di tale problematica perché si sottovaluta l'impatto negativo che l'incappare in questa situazione può provocare. Poiché più dei discorsi su questa materia servono i numeri, ho portato al Senato un solo esempio per far capire in quale spirale di incubo si entra a seguito di un furto di identità.

nel 2007, ancora oggi si trova a dover fronteggiare una situazione (e fornisco al riguardo numeri emblematici) che l'ha portata ad avere 33 assegni emessi a suo nome che hanno coinvolto otto banche, problemi con due carte di credito e 17 denunce per un importo totale di 266.410 euro. E non è ancora riuscita ad arrivare alla conclusione di questo megaequivoco (se così lo possiamo chiamare) nato nel 2007. Tutto comincia, per questa ed altre persone che subiscono furti di identità, con la sgradevole sensazione di trovarsi a chiedere un mutuo e scoprire di essere finiti in centrale rischi perché si era aperto, a propria insaputa, un foro nella propria identità; oppure di trovarsi ad avere assegni protestati o multe

25.000 casi di frodi creditizie. Rispetto all'anno precedente l'aumento è stato dell'11 per cento e si suppone che

Purtroppo il fenomeno si sta radicando. L'uso della strumentazione informatica infatti, diffondendosi, apre anche queste falle. A questo riguardo voglio richiamare l'attenzione dell'Aula su una problematica che è direttamente connessa con tale aspetto, vale a dire la necessità di

aiutarlo a non incorrere in queste frodi. Anche questo deve essere elemento di attenzione. L'uso degli strumenti informatici

Le frodi di questa natura sono agevolate dal fatto che non si fa un impiego corretto di alcune protezioni, quali l'uso del PIN dei propri telefoni o le modalità di modifica

dalla Comunità europea e dall'OCSE, che tendono a fare dell'educazione finanziaria uno strumento che possa entrare nei *curricula* scolastici per consentire di formare un cittadino consumatore che sia in grado di muoversi meglio all'interno delle problematiche che sempre più stanno diventando di interesse quotidiano nella vita delle persone e delle famiglie.

Il provvedimento che stiamo discutendo è certamente utile, completo e va approvato - ne convengo - in tempi assolutamente rapidi, ma poiché ci stiamo occupando di

Mi riferisco agli altri provvedimenti che riguardano il credito al consumo, pratica che sta diventando sempre più di uso quotidiano: sappiamo infatti che ormai si ricorre al credito al consumo per far fronte non a bisogni straordinari, ma a bisogni ordinari in momenti di crisi della vita delle famiglie. Si pone pertanto la complessa questione della capacità di autoregolamentazione delle proprie finanze e della capacità di leggere la gestione del proprio bilancio di leggere la gestione del proprio bilancio a fronte di indebitamenti delle famiglie che, attraverso il credito al consumo, si stanno facendo sempre più consistenti. Completare questo lavoro, anche in applicazione delle direttive comunitarie, significa occuparsi al più presto di credito al consumo pure in questa diversa accezione ed inoltre di educazione finanziaria, che è sicuramente lo strumento migliore per portare tutti i cittadini - di ogni età, ma soprattutto a partire dalle nuove generazioni che faranno sempre più i conti con strumenti informatici sofisticati - ad una capacità

portando al più presto all'attenzione dell'Aula anche i provvedimenti che ho richiamato. Il provvedimento in esame è assolutamente importante e diventa completo e non resta monco se attorno ad esso si costruisce una politica vera, concreta, non fatta soltanto di parole, di tutela del consumatore, che in questo momento di crisi è sicuramente un anello molto debole di una catena già di per sé fragile.

signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'argomento di cui stiamo discutendo è stato affrontato dalla Commissione finanze in sede referente, che ne ha concluso l'esame il 9 luglio 2009 conferendo all'unanimità alla relatrice Germontani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. La situazione generale del Paese, le difficoltà economiche delle famiglie italiane e il ricorso a forme di pagamento dilazionate o, comunque, differite nel tempo, rendono ormai indifferibile l'adozione di un organico intervento legislativo in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, nonché diretto a contrastare il reato del furto d'identità. La questione del furto di identità e della protezione dei consumatori e degli operatori nell'ambito delle attività che prevedono il pagamento differito ha assunto infatti dimensioni di grande rilevanza. La frode creditizia è un'attività criminale volta ad ottenere un credito o un bene con l'intento di non rimborsare il finanziamento o di non pagare quanto acquistato. Le frodi creditizie nel nostro Paese, attuate sia attraverso la sottrazione o la clonazione delle carte di credito sia tramite il furto d'identità, cioè il furto dei propri dati personali,

Le cronache recenti testimoniano la sempre maggior diffusione della pratica di procurarsi illegalmente informazioni personali e riservate con la finalità di ottenere illecitamente credito e acquistare beni o servizi, la quale costituisce ormai una vera e propria attività criminale organizzata.

Si tratta di un allarme serio, proveniente da una persona senza dubbio informata, dal momento che proprio Bernanke è rimasto vittima di un prelievo bancario effettuato da alcuni malviventi con l'utilizzo di dati sensibili della sua famiglia (la patente, che negli Stati Uniti sostituisce la carta di identità, il codice fiscale e le carte di credito). Trattandosi del Presidente della Fed, il lavoro dei servizi segreti e della polizia postale ha fatto sì che la rete delinquenziale venisse individuata e tratta in arresto. Ma non tutti i cittadini possono contare su tanta solerzia. È bene quindi che i malintenzionati abbiano ben chiaro il quadro delle sanzioni cui vanno incontro in caso di furto di identità, poiché senza una sanzione adeguatamente dissuasiva anche gli strumenti di prevenzione potrebbero rivelarsi armi spuntate. A tal fine proponiamo di inserire un articolo proponiamo di inserire un articolo 4-*bis* con il quale proponiamo modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il contrasto al furto d'identità.

ed il Governo. Vi è anche un altro problema, che riguarda le segnalazioni di insolvenza alla Centrale rischi della Banca d'Italia e ad altri sistemi di informazioni creditizie gestite da soggetti privati.

il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato il 1° aprile 2009 dal Gruppo IdV, con il quale si è impegnato ad adottare ogni utile iniziativa volta a garantire una piena tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento al cosiddetto diritto all'oblio degli interessati, assicurando l'applicazione uniforme delle determinazioni assunte dalle citate banche dati - soprattutto in relazione agli inadempimenti minori - con il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi; fare in modo che i nominativi dei cosiddetti cattivi pagatori (è l'altra faccia del furto di identità), ovvero di coloro che ritardano i pagamenti anche di pochi giorni o per modeste entità, vengano conservati nelle banche dati, con particolare riferimento a quelle private, per non più di tre anni dalla data di scadenza del contratto, al fine di non rendere difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente avesse provveduto a regolarizzare la sua posizione; fare in modo che le segnalazioni delle morosità nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali dei rischi e nelle altre banche dati, con particolare riferimento a quelle private, vengano effettuate solo in caso di mancati pagamenti di somme rilevanti, al fine di tutelare tutti coloro che, vedendosi rifiutare il credito da parte degli istituti finanziari, possono finire vittime dell'usura. Per fare in modo che il Governo tenga fede agli impegni presi con l'approvazione del citato ordine del giorno, abbiamo ritenuto utile presentare alcuni emendamenti al provvedimento in esame volti a tutelare i cittadini che si ritrovano iscritti e segnalati come insolventi sia nei sistemi creditizi gestiti dai privati sia alla Centrale dei rischi costituita presso la Banca d'Italia. Quest'ultimo è un sistema di raccolta nel quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti delle banche. Nel predetto archivio sono inseriti i dati di tutti coloro che risultano esposti con la banca per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamenti, cioè di coloro che vengono dichiarati insolventi. Situazione diversa è quella di coloro che vengono segnalati per esposizione superiore alla soglia di riferimento, anche se l'andamento del rapporto creditizio è regolare. In questi casi la concessione di nuovi crediti sarà approvata previa valutazione della solvibilità del richiedente. che per noi ha carattere di urgenza perché l'iscrizione nei sistemi di informazioni creditizie, nella centrale dei rischi e nelle altre banche dati, immotivata o conseguente ad erronee valutazioni o a segnalazioni di lievissima entità, in seguito alla quale colui che si rivolge ad una banca per avere un prestito si vede negare il credito, rappresenta l'anticamera dell'usura. Abbiamo già ricordato che ci sono sistemi di banche privati - come la CRIF - che vantano di aver schedato nelle proprie banche dati 50-60 milioni di posizioni, all'interno

destinata alle centrali rischi e agli istituti finanziari che aderiscono ai sistemi di informazioni creditizie, ai cui contenuti i soggetti interessati si sono dovuti attenere fin dal 15 dicembre Proprio per tutelare i cittadini che si ritrovano iscritti nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali dei rischi e nelle altre banche dati, immotivatamente o in conseguenza di erronee valutazioni o di segnalazioni di lievissima entità, abbiamo provveduto a presentare alcuni emendamenti che ci auguriamo vengano valutati

Per tale ragione auspichiamo che questi emendamenti che abbiamo presentato possano essere valutati con la migliore attenzione possibile. Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la Lega ha lavorato con impegno ed attenzione su questo provvedimento in Commissione insieme agli altri Gruppi in modo veramente fattivo e produttivo.

è che il sistema di acquisto dei beni e servizi con pagamento dilazionato e posticipato non interessa solo i cosiddetti beni durevoli, ma sempre più spesso anche quelli di consumo giornaliero, quali i generi alimentari, ed anche taluni servizi voluttuari, quali per esempio, quelli di cui

Queste due considerazioni, da sole, fanno capire l'opportunità e la necessità di un intervento legislativo in tale materia. L'intervento deve essere teso a dare maggiori garanzie ai vari soggetti coinvolti che sono ovviamente le banche, gli operatori finanziari, i venditori e i consumatori. Riteniamo assolutamente positivo il fatto che la proposta di legge, che è frutto anche di una sintesi proficua tra i due disegni di legge presentati dalla maggioranza e dall'opposizione su questo tema in Commissione,

costi. Altrettanto positiva è la specifica previsione che non ci debbano essere nuovi o maggiori costi a carico dello Stato, anche per i motivi che esponevo prima. Sarebbe importante garantire un'analoga assenza di nuovi o maggiori costi anche per i consumatori e le imprese che intendano procedere ad un acquisto con pagamento dilazionato e differito, mentre il sistema, in un certo senso, si sostiene

Signora Presidente, signor Sottosegretario, i due provvedimenti unificati al

dei colleghi, in un clima di collaborazione e con l'intendimento di raggiungere una piattaforma

ma perché questa convergenza incontra anche il consenso delle associazioni in questo caso interessate. Diamo un messaggio di fiducia. Nel piccolo questo provvedimento si inserisce all'interno di una grande problematica, quella che si è aperta con la crisi economico-finanziaria nella quale ancora ci dibattiamo e che poteva essere ancora più grave e drammatica se non fossero intervenuti subito elementi tesi a garantire fiducia e diretti a stabilizzare la crisi proprio dando ai consumatori e ai cittadini l'idea che la fiducia non veniva meno. Questo in termini macroeconomici ha significato - come ben sappiamo - il trasferimento massiccio

che impaurisce e rende meno stabile la convivenza civile; analogamente, in questo caso trattiamo di un problema che riguarda la sicurezza in una serie di attività, come quella del credito al consumo, appunto: se in essa manca un elemento di certezza, di stabilità e di fiducia, ciò provoca nel cittadino disorientamento e innesca una spirale davvero pericolosa.

cui l'introduzione dei sistemi di pagamento elettronici è avvenuta prima e dove il ricorso all'indebitamento anche per le piccole spese rappresenta una costante,

In questi giorni ovunque, sulla stampa, nei dibattiti, siamo portati a sottolineare questo grande elemento che campeggia nella riflessione sulla parte - speriamo conclusiva - della recessione e della crisi, vale a dire l'esigenza di fondare nuove regole, di ripristinare le regole nell'economia. Con questo

cerchiamo di dare l'idea di una regola che è prima di ogni altra attività. Il cittadino deve sapere che, se fa ricorso allo strumento del credito per il consumo, non è in balia dell'avventura. Lo abbiamo visto anche nella crescita portentosa e inaspettata del commercio per via elettronica: nessuno era fiducioso, soprattutto qui in Italia, che potesse esserci questa curva ascendente così accentuata e così rapida; invece c'è stata perché man mano che la fiducia è cresciuta e via via che il cittadino consumatore si è reso conto della plausibilità, della correttezza e, quindi, anche della comodità, in un regime di garanzia, di quello strumento, lo lo stesso è diventato di uso corrente e ha cominciato a rappresentare una possibilità per molti. Il modello di prevenzione e di monitoraggio richiede, come il disegno di legge ha previsto, strumenti di accertamento, innanzitutto; ma subito dopo si introducono elementi di deterrenza, perché non è possibile immaginare che noi stabiliamo l'idea che vi è una condizione di maggior tutela per il cittadino consumatore se accanto al monitoraggio e all'accertamento non vi sia anche una deterrenza. c'è l'esigenza, che viene contemplata nel provvedimento, di ridurre il contenzioso, perché molta parte del sovraccarico che vi è nell'attività amministrativa soprattutto delle società che operano in questo settore deriva da un contenzioso di difficile risoluzione proprio perché vi è ancora oggi molta incertezza e oscurità nelle procedure che poi portano alla frode. Credo, cari colleghi, che vada anche sottolineata, come hanno fatto coloro che mi hanno preceduto, la capacità che vi è stata di individuare un modo corretto per non realizzare una riforma piccola come questa, ma significativa caricando il bilancio dello Stato di altri oneri che, a fronte dei benefici, potrebbero essere facilmente contestabili. Questo modello di prevenzione e di monitoraggio, che fa capo all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento presso il Ministero dell'economia, è un sistema che, a giudizio dei colleghi che hanno lavorato particolarmente nella redazione del testo, non comporterà oneri eccessivi. Con il pagamento di una modestissima tassa di accesso, che ovviamente deve essere posta a carico dei fruitori, è possibile immaginare come la nostra previsione di un costo zero sia assicurata e certificata.

quindi, tra i Paesi virtuosi e non virtuosi al tempo stesso, ma certamente questo fenomeno della moneta virtuale e del ricorso al credito con strumenti di tipo elettronico sarà sempre più presente in futuro. Quindi, stiamo lavorando non solo per comprendere in che modo nell'immediato, adesso, oggi, si riesca a dare un segnale di stabilizzazione rispetto a queste procedure, ma guardiamo soprattutto al futuro e a ciò che avverrà in prospettiva.

con una parte in cui è possibile stipulare un'assicurazione, quale che sia, ad una tariffa contenuta e un'altra parte del Paese, peraltro più debole dal punto di vista del benessere e delle risorse, che paga il prezzo di una tariffa accentuata perché il fenomeno delle frodi è più diffuso.

e che sia significativo che l'opposizione abbia assicurato piena collaborazione e disponibilità nell'affrontare con rigore una materia così delicata come quella al

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione concerne problematiche che attanagliano il mondo del credito rendendolo insicuro soprattutto per coloro (gli utilizzatori finali, in massima parte persone fisiche) che hanno notevoli difficoltà a prevenire i rischi nello specifico settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e nel settore assicurativo (parlo degli indennizzi fraudolenti, eccetera), rischi connessi sia al furto di identità, sia a vere e proprie manovre fraudolente al fine di ottenere benefici per l'operatore (chiamiamolo così) disonesto. Ricordo che il furto d'identità (*identity theft*) è un meccanismo fraudolento, mediante cui un soggetto si appropria dei dati identificativi (nome, documento d'identità, numero della previdenza sociale o del Servizio sanitario nazionale, iscrizioni ad albi, carte di credito, eccetera) di altro soggetto (soprattutto persona fisica o anche giuridica) al fine di ottenere un ingiusto profitto. Il furto d'identità è quasi sempre operazione prodromica al compimento di fatti delittuosi che possono manifestarsi o nella clonazione di carte di credito (azione questa già soggetta a speciale vigilanza, in forza della legge 17 agosto 2005, n. 166) oppure (ed è il caso d'interesse del provvedimento in esame) con manovre illecite nel settore del credito al consumo. al consumo. Esemplificando, si tratta di attività, ovviamente illecite, volte ad ottenere un credito od un bene od un servizio con l'intento di non assolvere al pagamento relativo e con «accollo» della spesa al terzo ignaro dell'operazione,

effettua un acquisto a rate, ottenendo subito il bene o il servizio, ma caricandone il costo al soggetto di cui ha assunto l'identità. Ricordo che con l'espressione «credito al consumo», *ex* articolo 121, comma 1, del Testo unico bancario (TUB), si deve intendere «la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». I soggetti che possono esercitare tale attività, secondo il disposto dell'articolo 121, comma 2, del TUB, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, sono tutti gli imprenditori autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio dello Stato, nella sola forma però della dilazione del prezzo e non quindi della concessione del credito. Le frodi creditizie, come sinteticamente delineate, comportano rilevanti danni al nostro sistema economico: pur non toccando i vertici del mondo anglosassone, secondo i dati recentemente diffusi da un'agenzia preposta alla tutela dei consumatori, nell'anno 2007 sarebbero state rilevate ben 22.500 frodi, per un valore di oltre 110 milioni di euro. Il provvedimento oggi in discussione istituisce un sistema per prevenire gli illeciti di cui si è detto.

da notare che il citato ente opera già dal 1º gennaio 2008, per consentire il contrasto delle frodi nel settore delle carte di credito, di cui alla richiamata legge n. Possono aderire al costituendo nuovo archivio tutti i soggetti abilitati alla concessione del credito al consumo, i gestori di servizi di comunicazione elettronica, quelli di informazioni creditizie e le società di mediazione creditizia, soggetti tutti elencati all'articolo 1, comma 5, del provvedimento, nonché successivamente anche gli enti esercenti l'attività assicurativa. Tali soggetti potranno richiedere all'archivio la verifica dei dati indicati da colui che richiede la prestazione creditizia o assicurativa. Le richieste d'informazione comportano il pagamento di un corrispettivo, di importo tale da coprire - si spera - il costo dell'operazione, così da non gravare significativamente sul bilancio dello Stato. Le richieste promosse dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza non comportano alcun pagamento. Gli aderenti al sistema, inoltre, trasmetteranno all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode,

1'istituzione di un servizio telefonico e telematico assolutamente gratuito per il cittadino - ciò è molto importante - che potrà così segnalare le frodi subite o di cui teme di essere vittima. Verrà poi costituito un gruppo di lavoro, sempre sotto 1'egida dell'UCAMP, costituito dagli aderenti al sistema e da altri soggetti operanti nel settore con il compito di elaborare dati statistici (in forma anonima) delle frodi rilevate e di predisporre una relazione annuale al Ministero dell'economia e finanze che, sulla base di tali dati, riferirà al Parlamento. Per quanto concerne infine il settore assicurativo, l'articolo 7 del provvedimento prevede che con apposito decreto venga istituito successivamente un sistema di prevenzione per contrastare le frodi soprattutto per le richieste di risarcimento o indennizzo Si tratta di un provvedimento che, come già segnalato dalla relatrice, dopo un lungo *iter* iniziato nella precedente legislatura giunge in quest'Aula per la sua approvazione. Esso trae origine ed unifica due distinti disegni di legge proponendo un sistema di norme di tutta necessità che comporterà sicuri benefici per la nostra economia, senza eccessivi aggravio di costi per l'Erario,

Da ultimo, mi sia concesso esprimere il mio plauso per il lavoro svolto da tutti, e sottolineo tutti, i componenti della 6a Commissione permanente per far pervenire il provvedimento all'odierna seduta.

soprattutto per il lavoro concorde svolto in Commissione che credo abbia portato ad un risultato largamente condiviso.

Gli elementi comuni sono anche quelli relativi alle persone che mettono in atto queste frodi perché evidentemente chi può frodare nell'ambito delle carte di credito può farlo anche nella clonazione delle carte telefoniche così come nell'ambito delle assicurazioni. Avere questa banca dati diventa quindi l'elemento base per costruire una serie di interventi coordinati finalizzati a contrastare le frodi in questi ambiti.

Il provvedimento in esame non si pone l'obiettivo di risolvere singole e specifiche tipologie di frodi, ma vuole porre in essere elemento base volto a costituire un archivio, una banca dati, al quale i vari organi di sorveglianza, di vigilanza e investigativi, nonché le associazioni di categorie e le imprese interessate possano accedere al fine di evitare di incorrere in una determinata frode. Questo è l'obiettivo che si pone il provvedimento in esame e il Governo vorrebbe attenersi a questo stretto senza intervenire su una serie di altri argomenti che vanno ad inficiare norme di portata molto più vasta.

«La 1a Commissione permanente, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

2.500, 2.501 e 4.300 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

il quale prevede che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi di fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e - qui interviene l'emendamento - al Nucleo speciale di polizia

dopo il comma 2, intende invece rafforzare il dispositivo di prevenzione del furto d'identità e delle frodi nel settore del credito al consumo. consumo. A questo scopo il Ministero dell'economia, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni previste all'articolo 1, può avvalersi della collaborazione - e in questo senso va l'emendamento - del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 19 marzo 2001, attraverso l'utilizzo di strutture e personale esistenti

sia dal punto di vista del coinvolgimento delle competenze della Guardia di finanza, che sono assolutamente preziose in questa logica, sia ribadendo il principio (che in qualche modo attraversa

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, si possa aggiungere ogni altro dato idoneo -

al decreto iniziale attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, che in base all'articolo 6 deve essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

i costi economici riguardanti il pagamento del servizio dell'accesso alla banca dati non possono generare una traslazione sulle condizioni economiche degli utenti.

di sostituire le parole da «Al fine» fino a «assicurativi richiesti» con le seguenti parole: «i costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica dell'autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti».

il coordinamento riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, in cui è prevista una relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sulle frodi, a cui si allega anche la relazione da parte del Garante sul provvedimento in genere ma anche sul fatto che non vi siano le traslazioni di prezzo. Questo è il motivo della riformulazione. Se avessimo fatto un'integrale sostituzione del comma, sarebbe saltato il riferimento alla relazione del Garante.

non entra in contrasto con le indicazioni contenute in altri articoli; inoltre rappresenta un rafforzativo che qualifica ulteriormente la prima parte dell'emendamento, laddove si vincola al non effetto di ricaduta sugli utenti dei costi di funzionamento del sistema. Con il monitoraggio affidato ai meccanismi indicati ci auguriamo possa emergere l'esito che, se che, se si riduce l'area di rischio, anche i costi complessivi dei servizi diventano meno onerosi e, conseguentemente, anche gli utenti e i consumatori possono riceverne un beneficio. Sarebbe bello che il monitoraggio potesse certificare, non solo il rispetto della prima parte della norma, ma anche l'esito positivo di questo intervento.

od altri espedienti che permettono, impiegando i dati altrui, di ottenere dei guadagni illeciti con il credito o al consumo. Ci sono anche aspetti

delle spese di istruttoria o di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti, perché talvolta le formulazioni in cui questi valori vengono indicati nascondono aspetti nascondono aspetti fraudolenti nei confronti del consumatore. Nel nostro emendamento abbiamo anche illustrato altri elementi di correzione, alcuni citati anche in altri emendamenti, per quanto

eventualmente, l'implementazione di tali norme con altre più cogenti, ed in grado di essere più pregnanti, a favore del consumatore (che spesso sappiamo essere

la sempre maggior diffusione della pratica di procurarsi illegalmente informazioni personali e riservate con la finalità di ottenere illecitamente credito e acquistare beni o servizi. Tale pratica costituisce ormai una vera e propria attività criminale organizzata. L'utilizzo illecito di dati identificativi altrui è messo in pratica sia mediante strumenti tradizionali, quali furto della corrispondenza o dei documenti, che attraverso sofisticati, ma sempre più numerosi, stratagemmi di pirateria informatica. Il fenomeno, che fino a qualche tempo fa si riteneva apportare danni confinati alla dimensione finanziaria di singoli soggetti, ha raggiunto dimensioni tali da far ritenere che esso non provenga più, nei casi più eclatanti, da ambiti artigianali, quanto piuttosto da vere e proprie organizzazioni specializzate. Ho già ricordato che recentemente il presidente della *Federal Reserve* Bernanke ha dichiarato che: «Il furto di identità è un crimine serio», ricordando che colpisce milioni di americani. Che vi sia necessità di intervenire in materia, lo dimostra, dal lato tecnico, il fatto che a livello comunitario sono allo studio migliori sistemi di protezione degli utilizzatori della rete Internet, anch'essa esposta, come i più comuni documenti cartacei, alle insidie dei truffatori, la cui incidenza sulle transazioni, anche secondo i più recenti studi, sta acquistando preoccupante consistenza. Già la legge n. 547 del 1993 nacque sulla spinta di una raccomandazione del Consiglio d'Europa ed infatti, sin dal 1991, si è posta la necessità di norme a tutela delle carte di pagamento elettroniche. Numerosi sono gli accorgimenti che ciascuno può opportunamente adottare al fine di evitare e di ridurre la possibilità di cadere vittima di simili attività fraudolente. Significative in tal senso sono anche le norme approvate alla fine della scorsa legislatura in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Budapest nel novembre 2001. Le modifiche apportate alla legislazione vigente dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, hanno infatti prodotto un significativo affinamento degli strumenti giuridici nel settore dei crimini informatici. Ma resta pur sempre, segnalata dai giuristi informatici, la necessità di valutare la possibilità di un intervento più incisivo sugli aspetti penali della questione.

ed è operata con determinate modalità, non possa essere sanzionato meno duramente del furto. Sulla quantificazione della pena o sull'arricchimento/affinamento delle condotte tipiche si può aprire un dibattito utile, così come sulla collocazione sistematica del nuovo articolo nell'ambito del codice.

hanno bisogno del credito al consumo, vanno in un centro commerciale, fanno la richiesta (perché in tempi di dura crisi economica le disponibilità finanziarie si assottigliano)

maturato grazie al credito al consumo - che incide notevolmente sul proprio reddito residuo disponibile ed utile quindi al mantenimento della normale vita familiare. Molti

che, nell'ambito di quest'operazione finanziaria e di consumo, hanno un interesse affinché il sistema del credito al consumo sia sano.

i costi a carico dei consumatori sia i costi indiretti, nel caso venga meno la fiducia a questo strumento, a carico del mediatore finanziario o dei produttori. È importante rendersi conto che questo è un primo punto di partenza al quale dovranno seguire dei provvedimenti molto attenti affinché tutte le parti in gioco siano da un lato tutelate e dall'altro controllate in modo che tutto il sistema possa essere davvero un sistema di servizio agli scambi, alla crescita economica del nostro Paese e alla tutela dei consumatori.

si porta a conclusione un lavoro avviato già nella precedente legislatura e proseguito con un confronto approfondito in questo anno di nuova legislatura; si interviene su un tema delicato, un fenomeno assai diffuso e in via di progressiva espansione. Il furto d'identità è un'attività ovviamente illegale che inquina i rapporti tra soggetti erogatori e utenti facendo elevare il tasso di prudenza e di cautela con riflessi negativi verso i clienti e soprattutto danneggia chi ne resta inconsapevolmente vittima determinando disagi e costi di notevole portata. Con il disegno di legge che approveremo si afferma un modello di prevenzione fondato sul principio della razionalità, dell'essenzialità e della cooperazione. La banca dati, che è il perno di tutto il meccanismo, affidata alla gestione dell'UCAMP è un sistema flessibile; non costituisce nuove sovrastrutture di *hardware*; interconnette banche dati già esistenti e consente a queste di esprimersi al meglio in termini di funzionalità. Da questo punto di vista, anche per altri ambiti

Si rispettano, attraverso il meccanismo che è stato individuato, le norme della *privacy* avendo però contemporaneamente costruito un impianto che aiuterà davvero a prevenire il rischio di furti di identità e che permetterà anche, attraverso il monitoraggio impostato, di di osservazione e controllo di fenomeni anche nelle loro prevedibili evoluzioni in negativo, nel senso che anche chi agisce con il furto di identità non sta fermo, ma cerca sempre di aggirare i vincoli e le soglie di sbarramento che sono stati introdotti. Aggiungo ancora che si considerano molto importanti le attenzioni che sono state introdotte a beneficio dei consumatori, ai quali si riconosce una facoltà di interlocuzione e possibilità propositiva nel rapporto con il gruppo di lavoro che presidia l'intero sistema, e la relazione sull'andamento del fenomeno, soprattutto nella parte che coinvolge il cosiddetto *Mister* prezzi, che si prevede a salvaguardia del fatto che i costi di funzionamento non vengano traslati sugli utilizzatori. Io aggiungo e ribadisco che il nostro obiettivo è che l'efficienza che si conseguirà grazie a questo sistema e la riduzione dei costi che ne deriverà per tutti gli attori possano portare ad un abbattimento degli oneri a carico dei clienti utilizzatori. Questo è l'obiettivo più importante, insieme a quello della prevenzione e del contrasto ai comportamenti delittuosi, che il provvedimento determina. Aggiungo poi che una volta tanto si arriva abbastanza in tempo, nel senso che la Comunità europea proprio in queste settimane, nel corso dell'estate, ha registrato il crescere del fenomeno del furto d'identità e delle frodi conseguenti ed ha attivato una procedura per monitorare e verificare come i vari Stati membri stiano disciplinando queste fattispecie

sufficientemente adeguata ed attrezzata ad interloquire con l'evoluzione dei processi che si stanno determinando. Infine, sottolineo un aspetto che mi sta molto a cuore. Credo che si sia lavorato bene.

mi pare che questa sia un'ulteriore piccola dimostrazione, una sorta di cartina di tornasole, del fatto che quando il Parlamento viene messo in condizione di lavorare in maniera proficua l'opposizione reagisce e risponde in termini positivi e propositivi e che complessivamente l'istituzione nel suo complesso è in grado di produrre risultati legislativamente di qualità nell'interesse del sistema Paese. Se questa invece che essere un'eccezione, anzi un'estrema eccezione, potesse ridiventare la regola e la norma, credo che ne guadagnerebbero la democrazia e la funzionalità delle istituzioni nel nostro Paese.

avendo a questa materia lavorato non poco insieme al senatore Barbolini nel corso della passata e anche dell'attuale legislatura.

Quello del furto di identità e, in generale, delle frodi nel settore del credito al consumo e in quello assicurativo negli ultimi anni sono diventati problemi sempre più pressanti.

di crisi tanti italiani ed i problemi di liquidità che spingono ad un utilizzo crescente di forme di pagamento dilazionato. È appena il caso di dire che nel nostro Paese È appena il caso di dire che nel nostro Paese il comparto del credito al consumo è sensibilmente più contenuto rispetto ad altri Paesi ad economia avanzata, primi tra tutti quelli di lingua inglese e gli Stati Uniti d'America. Purtroppo, con la crescita del credito al consumo, tendono a crescere inevitabilmente anche il numero e la tipologia delle frodi nel settore dei finanziamenti, e non solo. Il diffondersi di certe frodi, peraltro, costituisce anche un costo improprio addossato agli operatori, nonché un onere assai gravoso a carico dei consumatori che ne restano vittime. Il testo sottoposto all'esame dell'Aula è stato oggetto di un approfondito dibattito in Commissione, grazie al quale il suo articolato è stato ulteriormente arricchito e perfezionato,

Esso origina da un lavoro di approfondimento compiuto nella precedente legislatura, come è già stato detto, visto che i due disegni di legge presentati inizialmente facevano riferimento ad un articolato già analizzato in 6ª Commissione. Nella presente legislatura tale lavoro è stato ripreso, in stretto contatto e collaborazione tra la Commissione finanze, il Governo e gli organismi che si occupano di vigilanza e del controllo su specifici settori, che vanno ringraziati per l'apporto che hanno fornito: mi riferisco in particolare alla Banca d'Italia, all'ISVAP, al Garante per la protezione dei dati personali e all'ANIA, l'Associazione delle compagnie di assicurazione, che a specifica richiesta sono state escluse dal novero degli enti che concorrono alla costruzione della banca dati, poiché in quella sede ne era già stata realizzata una di

Ad ulteriore dimostrazione di quanto il testo legislativo sia stato oggetto di approfondimenti, ricordo altresì il costruttivo apporto di tanti operatori del settore, volto a definirne meglio i contenuti e ad adeguarne le disposizioni rispetto alle esigenze che di volta in volta ci sono state segnalate. In questo senso, decisamente proficue si sono rivelate le audizioni svolte in sede informale in Commissione, poiché hanno visto coinvolti soggetti particolarmente qualificati, come ABI, Assofin, AISReC, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria e le organizzazioni dei consumatori e la Guardia di finanza. Ringrazio in questa sede anche la relatrice, come ho già fatto, per quanto si è spesa e per la proficuità della sua azione. In generale, si è riscontrato come sia particolarmente forte l'esigenza di operare efficacemente sul fronte amministrativo della prevenzione per limitare la portata del fenomeno, a supporto delle forze di polizia e del sistema giudiziario. In questa direzione, nell'ambito dell'Ufficio centrale antifrode sui mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si è prevista l'istituzione di un articolato sistema amministrativo di prevenzione delle frodi, composto da un archivio centrale informatizzato e da un gruppo di lavoro con la partecipazione di diversi soggetti. Concludo auspicando che una conclusione rapida dell'*iter* di questo provvedimento, come sta accadendo, possa consentire alla Camera dei deputati la definitiva approvazione. E per chi a momenti avesse ritenuto che questo provvedimento vada soltanto nella direzione di rimuovere l'occasione della frode, ricordo quanto Cesare Vivante, introducendo il capitolo dei titoli di credito nel nuovo digesto italiano, ebbe a dire: «A coloro che non sapessero cosa sono i titoli di credito dico subito che senza la cambiale e l'assegno non si sarebbe realizzata l'economia moderna». Questo del credito al consumo è un comparto

a chi concede credito al consumo di essere più predisposto, nell'esistenza di una chiarezza e di una trasparenza, alla concessione di maggiore credito foriero di sviluppo e di progresso come lo furono i titoli di credito ad avviso di Cesare Vivante.

e 507, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo»,

qualcosa che sta andando avanti dal febbraio 2008 è la certezza matematica che in questo Paese, da qualsiasi parte ci si giri, politicamente parlando, il rispetto della legalità costituzionale non viene praticato quotidianamente. La lettera è stata inviata al presidente Schifani, al Presidente della Camera e al Presidente della Commissione di vigilanza, dal segretario dell'Associazione Coscioni Marco Cappato, dal tesoriere Rocco Berardo, e dai copresidenti Maria Antonietta Farina Coscioni e Gilberto Corbellini. In Italia sono stati abrogati di fatto gli spazi di comunicazione riconosciuti dalla legge n. 103 del 1975, che prevedeva che ai partiti, ai Gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, a quelli nazionali, ai movimenti cooperativi giuridicamente riconosciuti nonché a gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta vengono consegnati degli spazi cosiddetti dell'accesso, che sono stati in parte, negli anni passati, concessi. Ebbene, tutto ciò ancora - ma mi è stata segnalata un'agenzia che lo smentirebbe - non è stato definito perché manca la creazione di una sottocommissione all'interno della Commissione di vigilanza RAI. Manca la Manca la sottocommissione perché, proprio come all'inizio di questa legislatura, mancava un accordo sul nome della persona che avrebbe dovuto presiederla. della Presidenza - che il presidente Zavoli abbia deciso di convocare a oltranza l'Ufficio di Presidenza per arrivare a questa elezione. Posto che la conferma, almeno sulle agenzie, non sono ancora riuscito a trovarla, questo è l'ultimo tassello di qualcosa che va avanti, per quanto riguarda questa legislatura, dal primo giorno: si mantiene l'Italia all'oscuro della possibilità di far circolare e conoscere le idee, ma allo stesso tempo si convocano gli italiani in piazza per la libertà di informazione sabato 19 settembre, con un silenzio assordante anche da parte della maggioranza, che pare in questo caso continui a non collaborare con la Presidenza della Commissione stessa per dare finalmente la possibilità alle associazioni di avere accesso alla RAI-TV. **Per

una nave con a bordo alcuni tecnici della Regione Calabria, su indicazione della procura della Repubblica di Paola, ha individuato, al largo delle coste tirreniche calabresi, un relitto con a bordo dei fusti di natura sospetta. Un'indagine immediatamente avviata ha dimostrato che si tratterebbe di traffico illecito di materiale radioattivo. La notizia è stata ripresa con grande enfasi dai mezzi di informazione (giornali nazionali, televisioni e quant'altro), destando, come lei immaginerà, una situazione di allarme sociale da non sottovalutare. Le chiedo di sollecitare il Ministro dell'ambiente, al quale peraltro nell'immediatezza abbiamo rivolto un'interrogazione parlamentare

Penso sia importante che anche il nostro Paese abbia una grande strategia industriale. In questa fase di crisi tutti i grandi Paesi

Signora Presidente, mi associo alla richiesta del collega Bevilacqua perché il Governo riferisca circa il ritrovamento annunciato